L'ordine del giorno reca la discussione della relazione informativa del senatore Li Gotti, delegato dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 135, comma 10, del Regolamento, sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura della custodia agli arresti domiciliari - ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, nonché degli articoli 4 e 5 della legge n. 140 del 2003 - decisa dal tribunale del riesame di Bari nei confronti del senatore Alberto Tedesco

Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo scorso 23 febbraio 2011 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari ha chiesto al Presidente del Senato l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Alberto Tedesco, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti. Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 24 febbraio 2011. Il successivo 7 marzo 2011 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta la documentazione integrativa inviata dall'autorità giudiziaria.

ascoltando il senatore Tedesco, ai sensi dell'articolo 135 del Regolamento. In data 8 marzo 2011 il senatore Tedesco ha depositato una memoria scritta allegando determinati atti, analiticamente elencati nella relazione scritta. Il 24 marzo 2011 la Giunta ha acquisito l'ordinanza del GIP con cui è stata respinta l'istanza di revoca della misura cautelare Il successivo 5 aprile 2011 il senatore Tedesco ha inviato copia della richiesta di archiviazione formulata dai pubblici ministeri di Bari nell'ambito del procedimento conclusosi con decreto con decreto di archiviazione emesso dal GIP, dottor Di Paola. L'ordinanza del GIP contenente la domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare indica gli elementi di colpevolezza ai sensi dell'articolo 273 del codice di procedura penale, e in essa sono indicate le esigenze cautelari ai sensi dell'articolo 274 L'ordinanza è stata adottata sulla base delle ipotesi di incolpazione relative ai reati di concussione, tentata concussione, concorso in tentata concussione, concorso in turbativa d'asta, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, concorso in abuso d'ufficio, falsità materiale e falsità ideologica. La richiesta del pubblico ministero faceva riferimento ad undici capi di incolpazione, ma il GIP ha accolto la misura limitatamente a sei capi di incolpazione. è stata rigettata dal GIP la richiesta di applicazione di misura cautelare per il più grave dei reati contestati, quello concernente l'associazione a delinquere. Il GIP, infatti, nella motivazione ha ritenuto che il sodalizio facente capo all'ex assessore Tedesco non possa essere assimilabile a un'organizzazione a delinquere «tenuto conto che in questo gruppo gran parte degli adepti non si conoscevano fra loro e alcuni (...) vi erano entrati non certo per dare un contributo al raggiungimento di non conosciuti né da loro conoscibili

il GIP ha recepito la richiesta della procura della Repubblica escludendo che ricorressero le ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso

le condizioni di cui alla lettera *c)* dello stesso articolo, ossia il pericolo di reiterazione delle condotte illecite. Nello stesso provvedimento motivazionale, il GIP ha esaminato gli elementi relativi al rischio di reiterazione, in modo particolare agli elementi soggettivi della personalità e al dato, che non può essere ovviamente pretermesso, riguardante la situazione soggettiva giuridica del senatore Tedesco, al quale venivano contestate ipotesi di reità riferite all'esercizio del suo mandato di assessore alla sanità della Regione Puglia,

Il GIP ha ritenuto che gli episodi contestati sono «maturati nell'ambito di un sistema incentrato essenzialmente su logiche clientelari di controllo del territorio», sistema nel quale l'ex assessore Tedesco avrebbe avuto «un indiscusso ruolo apicale». che tale ruolo non sarebbe correlato alla carica di assessore regionale, bensì alla «sua posizione di *leader* di una fazione politica inserita nella maggioranza di governo regionale». è un passaggio di particolare rilievo, ricavabile da alcune intercettazioni, citato nella motivazione dal GIP, ove è detto che da alcune intercettazioni si fa discendere in proposito che la qualità di senatore della Repubblica è «da considerarsi idonea a garantire, in via strumentale, la prosecuzione degli affari illeciti nel campo della gestione sanitaria». Rispetto a questa situazione, il senatore Tedesco - come dicevo poc'anzi - ha presentato una memoria scritta l'8 marzo 2011, il cui contenuto è articolato innanzitutto nella ricostruzione temporale dei suoi ruoli pubblici, ossia sul fatto d'aver egli presentato le dimissioni da assessore il 6 febbraio 2009, di aver continuato a far parte del Consiglio regionale per ulteriori cinque mesi, senza essere colpito da irrogazione di misure cautelari misure cautelari che - in quella situazione - non avrebbero avuto bisogno di alcuna autorizzazione, non essendo egli coperto da immunità. A suo avviso, proprio in ciò si potrebbe ravvisare un primo *vulnus* del procedimento, in considerazione del fatto che le indagini erano iniziate all'incirca nella prima metà del 2008, il che equivale a dire che per circa un anno e mezzo (marzo 2008-luglio 2009) non si era ritenuto necessario applicare misure cautelari, sia nel periodo di permanenza nelle funzioni di assessore sia durante quello di esercizio del

Un altro esempio significativo che il senatore Tedesco ha citato nel documento scritto, con documenti allegati, in ordine alla unidirezionalità delle indagini ravvisato nel fatto che la procura avrebbe omesso di dare corso ad una querela per diffamazione da lui presentata nei confronti del coordinatore regionale dell'IdV il 20 dicembre 2007. Entrando nel merito delle incolpazioni, il senatore Tedesco, quanto alla concussione, ha richiamato la disciplina vigente per precisare che la valutazione dei direttori generali - che sarebbe stata lo strumento della concussione - non è di competenza dell'assessore regionale. Altra circostanza indicata è che in tre anni di indagine gli inquirenti non hanno ritenuto mai di sottoporlo ad interrogatorio, con ciò negandogli la possibilità di offrire i necessari chiarimenti. Ulteriore circostanza afferente il tema del *fumus persecutionis* deriverebbe dall'esistenza di due procedimenti paralleli - con numerazioni ovviamente diverse - uno di competenza della Procura Procura distrettuale antimafia, l'altro della Procura ordinaria, ma con gli stessi pubblici ministeri, confluiti per la decisione a due diversi GIP. Per uno dei due procedimenti vi era la richiesta di archiviazione: era il procedimento che vedeva come indagato o iscritto nel registro delle notizie di reato il presidente della Regione, Vendola, quello per il quale siamo chiamati a decidere - aveva seguito altro destino, con la richiesta da parte dei pubblici ministeri di applicazione di misura cautelare per il senatore Tedesco e per altri numerosi indagati. Si segnalava altresì che gli episodi contestati erano distanziati notevolmente nel tempo, spaziando dal 2005 al 2008, sicché si trattava di singoli episodi non legati da un costrutto unitario, dal momento che lo stesso GIP aveva escluso i necessari indizi di colpevolezza dalla pur evidenziata associazione a delinquere. Il venir meno dell'ipotesi di associazione a giudizio del senatore Tedesco, elideva la possibilità di intravedere l'esistenza di quella rete di relazioni e di rapporti in forza della quale il GIP ritiene sussistente l'esigenza cautelare. Peraltro - precisava il senatore Tedesco - le sue immediate dimissioni dall'ufficio di assessore alle politiche della salute avrebbero, di fatto, reciso ogni suo collegamento con la sanità pugliese, oggi gestita da altro assessore.

viceversa, sull'altro procedimento, per il quale i pubblici ministeri avevano chiesto l'adozione delle misure, vi era un parziale accoglimento. Assume il senatore Tedesco che i comportamenti dei due procedimenti siano sovrapponibili,

Il contenuto della memoria depositata veniva confermato ed integrato dal senatore Tedesco nel corso della sua audizione innanzi alla Giunta. Anche sullo specifico passaggio dell'elemento costitutivo della concussione, reato trainante delle ipotesi recepite dal GIP, si faceva notare come dagli atti non vi sarebbe stata nessuna imposizione nella nomina di dirigenti di uffici, bensì esclusivamente dei suggerimenti. Un altro tema introdotto dal senatore Tedesco è quello relativo al possibile conflitto di interessi tra le sue funzioni di assessore e le attività economiche ed imprenditoriali svolte dai suoi familiari A tal proposito, egli comunicava alla Giunta che al momento della nomina ad assessore egli aveva deciso di chiedere ai suoi familiari di cedere le quote che detenevano in una società; e per un'altra società aveva indotto i propri figli a trasformare la ragione sociale (la società non si occupa più di commercializzazione diretta e produzione di materiale sanitario, ma di commercializzazione per per conto di terzi). Peraltro, le società erano state costituite alla fine degli anni Ottanta e il volume di affari era pari al 5-7 per cento dello specifico ramo d'impresa a livello regionale. Su questo scenario interveniva la relazione del senatore Balboni, nominato relatore. Nella relazione proposta alla Giunta il senatore Balboni si soffermava inizialmente sul tema del dedotto *fumus* *persecutionis* analizzando le argomentazioni addotte dal senatore Tedesco e giungendo alla conclusione dell'insussistenza del *fumus* *persecutionis*.

da giustificare l'alterazione della piena funzionalità degli organi parlamentari derivante dalla modificazione del *plenum* assembleare a seguito dell'adozione di misura cautelare. Il relatore Balboni poneva in evidenza come, nel caso di specie, si tratti del bilanciamento di principi entrambi tutelati dalla Costituzione (ossia, di valutare il rispetto del principio dell'integrità del *plenum* nei confronti del principio dell'esercizio della giurisdizione con l'applicazione di misura cautelare),

concesso l'autorizzazione all'arresto di un suo componente. Vi sono dei precedenti che riguardano l'altro ramo del Parlamento, ossia la Camera, che ha in altri casi deliberato in senso positivo, ma con riferimento ad ipotesi di reati gravissimi come l'omicidio o la partecipazione a banda armata. Sulla base di questa impostazione, il relatore Balboni proponeva alla Giunta di escludere la sussistenza del *fumus* *persecutionis* e di valutare invece la salvezza del principio del rispetto dell'integrità del *plenum* assembleare rispetto ai reati, giungendo a una ponderazione degli interessi entrambi costituzionalmente protetti, ma sottolineando il prevalere del principio delrispetto *plenum* assembleare. In Giunta si sviluppava un'articolata discussione. Alcuni componenti della Giunta hanno ritenuto che non si fosse raggiunta con compiutezza la prova della inesistenza del *fumus* *persecutionis*, sicché sarebbe stato opportuno attendere l'esito del ricorso in appello proposto dal senatore Tedesco (ricorso che quando si svolgeva questa discussione in Giunta era pendente); si si consigliava pertanto di attendere tale esito prima di prendere la decisione. Quanto alla disparità di trattamento in quei due procedimenti paralleli, con esito diverso, di cui poc'anzi ho parlato (uno conclusosi con l'archiviazione e l'altro con l'adozione di richiesta di misura cautelare), la Giunta procedeva a valutare la consistenza dell'argomentazione

poteva configurarsi questa critica, non per le altre. Per quanto riguarda la linea del *fumus persecutionis*, indubbiamente in linea generale la Giunta era orientata ad affermare il principio che comunque il Senato non deve approcciarsi ad una valutazione di merito degli elementi probatori raccolti. Bisogna quindi mantenere una netta distinzione tra i diversi ambiti di competenza, evitando sovrapposizioni e condizionamenti. Un primo orientamento della Giunta, espresso da alcuni componenti, era quello secondo cui la valutazione doveva limitarsi a verificare la sussistenza o meno del *fumus persecutionis*. Il secondo orientamento era invece quello di verificare anche la gravità dei reati come elemento da ponderare rispetto al principio dell'integrità del *plenum* assembleare. La relazione del senatore Balboni non veniva approvata dalla Giunta, ma la varietà delle argomentazioni espresse dai diversi componenti non consentiva di fare emergere una relazione alternativa sicché, sulla base di questo risultato, la Giunta deliberava di affidare ad un suo componente una relazione meramente tecnica e senza conclusioni sulla vicenda.

l'ordinanza del tribunale del riesame, che era confermativa della misura cautelare ma con diverse modalità. In sostanza, non una misura cautelare in carcere, bensì una misura cautelare con arresti domiciliari. momento che la Giunta ha ritenuto che il titolo della misura cautelare non veniva scalfito dalle motivazioni del tribunale del riesame, ma si modificava esclusivamente la modalità dell'applicazione della misura, si è ritenuto esclusivamente di integrare questa relazione con tale dato oggettivo, ma di non mutare i contenuti giuridici della relazione stessa.

intervengo sull'ordine dei lavori, perché c'è qualcosa che io non ho compreso e che la relazione (se così possiamo chiamarla) del senatore Li Gotti non ha chiarito. Si tratta di questo: ha esaminato la relazione del relatore, senatore Balboni, e poi l'ha votata respingendola. La Giunta, però, non ha ritenuto che l'aver respinto la relazione Balboni equivalesse automaticamente all'approvazione di una relazione contraria.

perché la Giunta non ha votato la relazione contraria? Perché la Giunta non ha proposto la relazione contraria e non l'ha messa in votazione? E perché, per la prima volta nella storia del Senato, signor Presidente, noi ci ritroviamo una relazione senza relatore? Vede, signor Presidente, tra qualche minuto, o tra qualche ora, noi potremmo essere chiamati a dare un voto, e io non so se sarò chiamato a dare un voto sulla relazione Balboni, se saremo chiamati a votare la relazione del GIP o se saremo chiamati, peggio ancora, a votare la relazione del senatore Li Gotti, che non era ovviamente una relazione. Questo a me pare veramente cavilloso dal punto di vista della procedura che che assume il Senato. Mi chiedo perciò, signor Presidente, se lei non voglia chiedere conto al Presidente della Giunta, che mi sarei aspettato intervenisse prima del senatore Li Gotti, di questa strana procedura, perché se respingere una relazione non equivale (e su questo punto seguo) ad approvare la relazione contraria, perché allora non approvare la relazione contraria? C'è qualcosa di poco trasparente nella procedura di questa seduta, signor Presidente, così come c'è stato qualcosa, a mio avviso, di poco trasparente nell'andamento dei lavori della Giunta delle elezioni Poi ho visto ovviamente che alla fine ci siamo ridotti a richiamare l'articolo 135, comma 10, del Regolamento, il quale dice che certamente qualcuno della Commissione può venire in Aula, chi è venuto in Aula ha fatto una relazione esattamente come se fosse stato il vero relatore portatore di una relazione, invece il senatore Li Gotti non è venuto in Aula dicendo quello che mi sarei aspettato che lui dicesse, perché non ha preso una posizione, perché qui nessuno viene con una posizione.

Questo «in difetto» lascia presupporre che si possa ipotizzare la situazione nella quale ci troviamo, cioè che la Giunta non deliberi e che quindi in questo difetto di deliberazione della Giunta si voti in Aula la richiesta di autorizzazione.

vorrei far presente al senatore Pera che talvolta è cavillosa la situazione e non la procedura. Noi abbiamo seguito una strada di una certa linearità. In Giunta si era affidata la relazione al senatore Balboni, il quale ha formulato una proposta che non è stata approvata. La maggioranza La maggioranza che ha votato contro la proposta del senatore Balboni non era detentrice di una proposta diversa; anzi, all'interno di questa maggioranza - per così dire - c'erano ragioni diverse ed antitetiche. Per evitare di prolungare il lavoro della Giunta in modo artificioso, il Presidente della stessa, con il conforto di tutti i Gruppi presenti in Giunta, ha ritenuto di portare direttamente in Aula, secondo il Regolamento, non una proposta, sulla quale c'era una difficoltà politica a formare una maggioranza,

Questa è la situazione per quanto riguarda le decisioni che nella Giunta sono state assunte con il consenso di tutti i Gruppi, ovviamente tenendo informata la

Signor Presidente, colleghi senatori, innanzitutto intendo rappresentare all'Assemblea il mio sincero rammarico per il coinvolgimento in una vicenda che appartiene alla mia pregressa attività di amministratore regionale

ci hanno informati dell'indagine, ho immediatamente ed irrevocabilmente rassegnato le mie dimissioni da assessore regionale alle politiche della salute della Puglia. Sono veramente rammaricato per il fatto di dover costringere il Senato, peraltro nella nella coda dei lavori che precedono le ferie estive, ad occuparsi di tale questione. Tuttavia voglio ringraziare elezioni e delle immunità parlamentari e il suo Presidente per la possibilità che mi è stata concessa di esprimere compiutamente le valutazioni su quella richiesta che oggi occupa i nostri lavori, per aver potuto fornire alla Giunta in più circostanze chiarimenti che io ritengo dettagliati sulla vicenda stessa e quindi per avermi consentito direi una difesa appropriata di ragioni non pretestuose. In questa sede ribadisco la mia estraneità ai fatti che mi vengono contestati e addirittura contesto che esistano dei fatti penalmente rilevanti, trovandomi in buona compagnia in questa contestazione degli stessi PM che hanno chiesto il mio arresto: infatti, come è stato egregiamente illustrato dal collega Li Gotti, in un procedimento parallelo questi chiedevano l'archiviazione per alcuni fatti identici o per fatti sovrapponibili. in buona compagnia, inoltre, rispetto ad un GIP del tribunale di Bari che accoglieva quella richiesta di archiviazione, riteneva insussistenti come reato fatti che venivano etichettati, ascritti alla categoria dell'avvicendamento nelle nomine, fatti che addirittura venivano ritenuti penalmente non rilevanti in relazione persino alle nomine dei primari, dove quel GIP riteneva che un amministratore regionale ben poteva intervenire nella nomina dei primari, se questo intervento stato finalizzato a preservare il buon andamento del Servizio sanitario. Le vicende le conosciamo. Devo ringraziare sentitamente il senatore Li Gotti per la chiarezza espositiva di una relazione ricognitiva, e voglio rassicurare il senatore Pera che in questa sede esprimo le mie opinioni senza alcun vincolo e senza che alcuna pressione, né psicologica, né politica, sia stata esercitata nei confronti del sottoscritto. Anzi, denuncio come fantasiose quelle illazioni che ho letto veramente stupito questa mattina sulle pagine della rassegna stampa che vorrebbero attribuire ad un autorevole esponente del Partito Democratico una sorta di coercizione psicologica. Non sento quell'esponente da oltre sei mesi, né credo che sia nello stile di quel dirigente del mio partito esercitare pressioni di questo genere. Devo prendere atto, e lo faccio con qualche rammarico ma - devo dire - anche in questo caso con molta serenità, del fatto che la Giunta delle elezione e delle immunità parlamentari si è divisa sulle conclusioni alle quali sarebbe dovuta pervenire. Si è divisa con un voto negativo rispetto alla relazione del relatore di maggioranza che proponeva di non considerare positivamente la sussistenza del *fumus persecutionis* e, tuttavia, proponeva di tuttavia, proponeva di respingere la domanda della magistratura barese in relazione alla lesione di prerogative parlamentari non meglio precisate. In quella sede si sarebbero potuti, forse, meglio approfondire gli elementi che la magistratura ha portato all'esame di quest'organo, gli elementi che io stesso ho portato all'esame dello stesso organo. Tuttavia, rispetto assolutamente, come è doveroso fare, le conclusioni alle quali la Giunta è pervenuta rimettendo all'Aula, che in ordine a queste decisioni è sovrana ed ha competenza esclusiva, la decisione definitiva su questa vicenda. Fino a qualche giorno fa ero estremamente convinto di sostenere fino in fondo le ragioni della sussistenza del *fumus persecutionis*, e lo facevo, appunto, avendo maturato autonomamente questo convincimento. Tuttavia, le vicende che stanno caratterizzando la cronaca politica e che occupano, io credo, non solo le coscienze dei cittadini ma le coscienze degli addetti ai lavori della politica, delle istituzioni che li ospitano dovrebbero portarci ad una riflessione supplementare rispetto ad una valutazione che che rischierebbe di diventare burocratica se non si attingesse a categorie più profonde. Bisogna cioè assolutamente sanare questa sorta di cortocircuito che sta caratterizzando il rapporto la società italiana e le istituzioni che la rappresentano, un cortocircuito che va ascritto sicuramente ad una una superficiale valutazione dell'importanza di questo rapporto e anche, credo onestamente, ad una

Ma tant'è: oggi il Paese non si fida più delle proprie istituzioni. Siamo di fronte ad una condizione di emergenza, che non può essere derubricata alla stregua di una pur legittima difesa di prerogative costituzionalmente garantite. quindi che, pur potendo ulteriormente rivendicare un approfondimento di quest'Aula sulle tematiche relative al *fumus* *persecutionis*, oggi una valutazione di opportunità e la preoccupazione di farsi carico del valore profondo della funzione di rappresentanza di questa istituzione debba portarci a nemmeno adombrare il dubbio che in favore di qualcuno di noi si assuma un atteggiamento

è una cosa assolutamente intollerabile, che non può essere avallata da comportamenti che siano meno che trasparenti, meno che lineari,

colgo questa occasione, approfitto di questa opportunità che mi viene conferita dalla mia funzione parlamentare per sollecitare la magistratura ad intraprendere rapidamente la strada del processo. Il procuratore della Repubblica di Bari ha dichiarato due mesi fa che le indagini che mi riguardavano erano concluse, quindi francamente non si capisce per quale motivo, a distanza di due mesi, egli non abbia ancora adottato il relativo decreto di conclusione delle indagini, che aprirebbe la strada alla celebrazione di un processo. Allora, bisogna sgombrare il campo da tutti gli inceppi, a cominciare da quelli - sia pure apparenti - che costruiremmo se in quest'Aula ci opponessimo alla domanda della magistratura barese. Io credo che dovremo apertamente, in maniera trasparente, votare affermativamente rispetto a quella domanda.

sforzandoci di realizzare sulla questione l'unanimità di questo ramo del Parlamento, nella consapevolezza che probabilmente oggi rinunciamo ad un pezzo di un qualche nostro diritto, ma sapendo che questo diritto potrà risaltare sicuramente più forte nel momento in cui il cammino di una corretta gestione di una vicenda processuale si sarà concluso. Colleghi del Senato, se posso permettermi, io vi chiedo sommessamente ma fermamente di rispondere positivamente alla domanda della magistratura barese, di farlo alla luce del sole, offrendo le nostre facce come risposta di ciascuno a quella domanda. Concludo - se mi è consentito - con la frase di un esponente politico la cui memoria mi è molto cara, e che credo lo sia alla maggior parte dei cittadini italiani che hanno superato una certa età. Diceva Pietro Nenni: «Si faccia quel che si deve, accada quello che può». Credo che noi dobbiamo fare quello che si deve, e accadrà quello che potrà accadere, ma io sono convinto che accadrà quello che sarà giusto che accada.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non tocca a noi oggi sostituirci al giudice penale nel giudicare il collega Tedesco per i reati a lui ascritti. Questo però non ci esime dal dovere di esprimere un chiaro giudizio politico sul governo della sanità nella Regione Puglia, di cui Tedesco è stato per tre, devastanti anni, assessore, con l'aggravante della competenza, vista la sua antica dimestichezza del settore per ragioni sia politiche, di amministratore regionale di lunghissimo corso, sia di interesse personale e familiare. Negli anni di Tedesco la sanità pugliese, consegnata dal precedente governo di centrodestra con un attivo, documentato dai suoi stessi successori, di 9 milioni di euro e con un piano di ristrutturazione che l'avrebbe messa al sicuro nei conti ottimizzandone la qualità, è sprofondata sempre più in un baratro di opacità amministrativa e di dequalificazione dei servizi che, per la rapidità della sua evoluzione, forse non ha eguali in Italia, nell'assenza, non meno grave, di ogni programmazione. Certo è che, da una condizione di accertata virtuosità, essa è arrivata al punto di necessitare di un piano di rientro «lacrime e sangue», senza il quale - come riconosciuto dal suo stesso assessore al bilancio la Regione Puglia sarebbe precipitata in condizioni devastanti di *default*. La spiegazione di tutto questo è nelle carte dell'inchiesta a carico del collega Tedesco, che ci rappresentano il quadro angosciante di un autentico assalto alla diligenza, un saccheggio spregiudicato nel segno della totale occupazione della sanità da parte della politica, che si spingeva con i suoi tentacoli fino all'ultimo ripostiglio ed all'ultima seggiola disponibile e, quando non ve n'erano più, le moltiplicava per occupare anche quelle. mentre venivano artatamente azzerati tutti i controlli sulla spesa, pur di poter spendere senza controlli, ed i bilanci regionali saltavano l'uno dopo l'altro per effetto di sforamenti continui dei conti della sanità, fino a determinare tre sfondamenti del patto di stabilità in quattro anni, le liste di attesa per i cittadini pugliesi bisognosi di cure sanitarie si allungavano all'infinito, gli ospedali si riducevano a lazzaretti, i casi di malasanità divenivano la norma, fino a non fare più notizia. A conferma di quale fosse l'andazzo di quegli anni, basta leggere la stampa locale del 15 settembre 2005, che dava conto della spartizione capillare delle spoglie della sanità pugliese, che non si limitava all'assegnazione a partiti e partitini delle direzioni generali, ma si spingeva senza alcun pudore anche a quelle delle direzioni sanitarie ed amministrative, in palese violazione della legge che assegna tali scelte ai direttori generali, per scendere di fatto fino all'ultimo portantino, financo ad una bibliotecaria. Di tutto questo però sarebbe ingiusto incolpare il solo assessore, che peraltro era espressione di una sorta di suo partitino personale che non si vede come potesse avere da solo il monopolio dell'85 per cento del bilancio di una Regione in cui imperversavano, oltre a Vendola e ai vendoliani, i DS e la Margherita, poi confluiti nel PD. Ed infatti basta tornare a leggere le carte dell'inchiesta per vedere che a mal governare la sanità pugliese Tedesco non era affatto solo. È anzi assolutamente acclarato, anche dalla richiesta di custodia cautelare pervenutaci dal GIP De Benedictis, che di ciò di cui egli viene accusato quantomeno il governatore Vendola era informato e partecipe, salvo vedersi miracolosamente gratificare di un salvacondotto francamente inspiegabile, se non con l'antica regola per cui il pesce piccolo paga anche per il pesce grande. Una politica del doppiopesismo, spesso utilizzata da una parte della magistratura barese anche in altre vicende su cui tuttora gravano pesanti pesanti perplessità di terzietà di giudizio. Certo è che i baratri finanziari apertisi all'improvviso sotto la sanità pugliese ai tempi di Tedesco si sono riprodotti tali e quali anche senza Tedesco, con al suo posto il commissario politico che Vendola gli aveva imposto fin dal primo giorno, e che le lottizzazioni continuano ancor oggi, con un con un ex consigliere regionale DS e un candidato di SEL al Comune di Vicenza nominati alla guida delle due ASL più importanti di Puglia, in attesa di spartirsi tutto il resto. Né si può dire che Vendola non conoscesse il conflitto d'interessi che appesantiva il suo assessore. Al contrario, qualora già non lo conoscesse, ne era stato pubblicamente informato all'atto della nomina del suo governo e ne aveva avuto conferma pubblica dallo stesso interessato quando, nell'ottobre del 2007, l'argomento approdò in Consiglio regionale in un dibattito assolutamente franco che il Governatore concluse confermando platealmente la sua fiducia all'assessore, che aveva correttamente rimesso nelle sue mani il mandato. La verità è che Tedesco era l'ideale per il Governatore alla guida della sanità, sia perché sapeva dove e come metterci le mani, sia perché, come eventuale capro espiatorio, era pur sempre un povero socialista. ciò si evince chiaramente dai Resoconti anche della Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale del Senato, con riferimento in particolare alle audizioni di Vendola e dell'ex dirigente generale della ASL di Bari Cosentino. La prova definitiva del fatto che egli aveva molti crediti da incassare l'ha data il suo provvidenziale ingresso al Senato, con apposita liberazione del posto tramite il Parlamento europeo, a seguito di una campagna elettorale in cui Vendola, pur formalmente sostenendo un altro partito, lo aveva scortato più o meno dappertutto. Detto questo, non si può non rilevare che una richiesta di custodia di custodia cautelare che arriva dopo anni dai fatti contestati, in assenza ormai di ogni pericolo di reiterazione del reato, inquinamento delle prove o fuga, apparirebbe inspiegabile per qualsiasi cittadino. Si ha l'impressione quindi che la magistratura non abbia voluto perseguitare Tedesco, ma forse assolvere Vendola. Trattandosi di un parlamentare, fermo restando che egli non può e non deve sottrarsi al processo e alle sue conseguenze, essa si configura anche come una lesione della sovranità popolare, di cui ognuno di noi è espressione e depositario. Di qui il nostro voto, che non intende assolvere né Tedesco né tanto meno i suoi amici politici, ma confermare una cultura di garanzie, irrinunciabile presupposto di rispetto per quest'Aula, consentendogli di continuare ad esercitare il mandato che gli è stato affidato.

Io penso che noi siamo chiamati in questo momento a discutere di ben altro, e gli interventi dovrebbero essere...

perché non è questo il modo di comportarsi! Presidente, io mi permetto di ritornare sull'argomento sollevato dal senatore Pera.

il quale, in buona sostanza, solo in un caso la Giunta non si pronuncia, ossia quando il Ministro dà comunicazione che il relativo procedimento è cessato.

Attenzione, perché stiamo intervenendo su una questione che non riguarda un arzigogolo procedimentale, bensì un'attribuzione della responsabilità e dei ruoli, e tutti devono sapersi assumere le responsabilità!

la relazione del senatore Li Gotti sul punto del *fumus persecutionis*.

preliminari di custodia cautelare in carcere, che è stata invece modificata dal giudice superiore dell'impugnazione in arresti domiciliari. Ebbene, a me pare che questa modifica di fatto non sia indifferente; anzi, sia molto importante per verificare il *fumus* *persecutionis*. Com'è noto, le misure coercitive sono cinque, di gradazione successiva verso la più grave: il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l'obbligo o il divieto di dimora, gli arresti domiciliari e la custodia cautelare in carcere. Oso osservare una banalità: tre di queste, le meno gravi, sono tra l'altro compatibili con l'esercizio della funzione di deputato o senatore. Il divieto di espatrio consente di essere presente al Senato o alla Camera, così come l'obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria e l'obbligo o il divieto di dimora, perché se l'obbligo di dimora è a Roma, il senatore, nel caso di specie, potrebbe esercitare quelle funzioni che gli sono demandate. Allora, noi abbiamo una decisione della magistratura, quella del tribunale del riesame, secondo secondo cui la decisione del giudice delle indagini preliminari è stata sbagliata perché era sufficiente, per le garanzie che sono note della giustizia, la minore sanzione degli arresti domiciliari. Ma lo dice la magistratura, non lo diciamo noi: lo abbiamo soltanto ricordato. Ebbene, ciò vuol dire che la decisione del giudice per le indagini preliminari era sbagliata oggettivamente in riferimento a quanto aveva deciso, cioè la massima misura coercitiva.

cioè una misura coercitiva, che è una sanzione nei confronti del Senato), ma anche sul contenuto di questa richiesta.

dopo la decisione del tribunale del riesame, che ha dichiarato oggettivamente che la decisione del giudice per le indagini preliminari è in violazione pacifica dell'articolo 275, terzo comma, del codice di procedura penale, a tenore del quale, com'è noto, la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. L'avere obiettivamente errato da parte del giudice per le indagini preliminari su questo punto, oggettivamente errato, indipendentemente dalla volontà di un *fumus* *persecutionis*, realizza, secondo me, allo stato attuale, una non modesta prospettazione di *fumus persecutionis*, secondo quanto la stessa magistratura ha implicitamente ma significativamente detto.

può mancare la deliberazione è intimamente connessa alle condizioni previste dal comma 2. Se il Ministro, cioè, ha dato comunicazione della cessazione del procedimento, allora l'*iter* procedurale si deve concludere in Aula con una deliberazione dell'Assemblea. Quindi, non è possibile assolutamente che l'Assemblea si trovi a deliberare se sia carente il presupposto ipotizzato dall'articolo 2. Valentino, il Presidente si è già pronunziato su questo, e non intende rivedere la sua posizione, anche perché non può imporre ad una Giunta di pronunziarsi. Per analogia, abbiamo tanti esempi di Commissioni che non completano il proprio lavoro,

Non intendo indietreggiare su questa posizione, cioè di imporre alla Giunta un pronunciamento. Non è nei poteri del Presidente, perché, se così fosse, rischieremmo di essere paralizzati nel pronunziarci su una richiesta della magistratura. Questo - a mio avviso e secondo i principi dell'ordinamento giuridico e costituzionale - è impossibile.

Aveva la possibilità - e ce l'ha ancora - di dimettersi da parlamentare e di difendersi nelle sedi giudiziarie, così come ha fatto quando si è dimesso da assessore regionale. Giustamente, nella sua memoria difensiva, ha dato atto ai magistrati di nella sua memoria difensiva, ha dato atto ai magistrati di aver seguito due percorsi diversi. In un'intervista a "il Giornale", si legge: «Tedesco sfida Vendola: "Perché io sono in cella? Lui è un privilegiato"». Colleghi, il processo parte da un unico fatto: da un'associazione a delinquere costituita dal senatore Tedesco con altri otto personaggi che si muovono nell'ambito della sanità pugliese; si arriva a 11 capi di imputazione. Il senatore Tedesco, allo stato, è imputato per 11 reati, che vanno dall'associazione a delinquere,

solo quattro: la concussione, la tentata concussione, il falso e altri reati. È vero quando lei dice che i magistrati pugliesi hanno usato una doppia misura, nel senso che Vendola è stato archiviato lo stesso procedimento mentre lei oggi si trova sottoposto a giudizio. Come Gruppo di Coesione Nazionale siamo contrari all'arresto, signor Presidente.

stanno in carcere per aver commesso reati meno gravi, e vi sono stati pubblici amministratori o pubblici dipendenti sospesi dalle proprie funzioni per reati meno gravi. Caro senatore Tedesco, lei è un privilegiato. Le nostre condizioni in quest'Aula...

La scelta che il mio Gruppo ha operato è quella di attenersi al rigoroso rispetto delle norme, senza scendere ad un livello di polemica politica che porterebbe lontano. Alcuni colleghi hanno voluto fare ciò,

funzionari pubblici e con società di Alberto Tedesco e Gianpaolo Tarantini, conoscenza del *Premier* e fornitore del prodotto di cui il *Premier* era l'utilizzatore finale. sodalizio societario ben descritto nei provvedimenti, che hanno evidenziato come le conversazioni intercettate, già all'epoca, nel 2001, facevano emergere l'intento da parte di Tarantini e di Giuseppe Tedesco di dividersi il mercato regionale per aree commerciali. Questo è lo scenario politico. Quindi, abbandoniamo questa deriva, torniamo alla tecnica, perché la deriva ha bisogno di profeti più accreditabili.

Se ogni imputato del PdL dovesse procedere alle dimissioni, si arriverebbe allo scioglimento delle Camere per mancanza del numero legale. Avremmo risolto il problema dei costi della politica:

Voglio fare un discorso tecnico, ma purtroppo ci sono orecchie non aduse a questo linguaggio, e allora l'opzione che offro l'opzione che offro è quella di non ascoltarmi. Io non intendo essere ascoltato, gradisco anche le persone che non mi ascoltano. allora la nostra posizione? Apprezziamo il gesto di dignità del senatore Tedesco, che ha affermato di poter coltivare la tesi da lui sostenuta del *fumus persecutionis*, e però di aver deciso di rinunziare, considerando e valutando il particolare momento del Paese. Riteniamo che, nel caso in esame, non sussista il *fumus persecutionis*, né oggettivo, né soggettivo e, sgomberato il campo da questo profilo, noi non riteniamo che tecnicamente possa il Senato entrare nel merito delle accuse ipotizzate:

un giudice superiore dice che ciò si può ottenere con gli arresti domiciliari in casa. E vero, non è vero, è possibile? Questo è quanto prescrive il nostro codice, e non lo si può cambiare in questa sede. Dobbiamo fermarci

Rispetto ai due principi costituzionali, cioè l'integrità del *plenum* e l'esercizio della giurisdizione, qual è il valore che deve prevalere? Il senatore Balboni proponeva di valutare il peso dei reati per poi ponderarlo con il principio dell'integrità del *plenum*. Faccio presente che,

come Senato non possiamo assumerci la responsabilità di creare la condizione per la reiterazione delle condotte illecite. Questo è quanto prevede il giudice. Dunque, rispetto al principio della salvaguardia del *plenum* assembleare ritengo che debba essere ponderato anche l'ulteriore principio dell'impedire ciò che il giudice il tribunale del riesame hanno ritenuto essere concreto come fatto, ossia la reiterazione del reato. Di fronte a questo, tra i due interessi in ponderazione, riteniamo che prevalga

assolutamente condivisa e, pur con le riserve di fondo sull'istituto della misura cautelare, mie personali, sarà favorevole alla richiesta di concessione dell'autorizzazione alla misura cautelare.

Seguiremo le sue indicazioni votando a favore della richiesta dell'autorità giudiziaria. Pertanto, annunciamo il voto favorevole da parte del

e di cui rispettiamo da sempre l'operato, lontani peraltro da ogni forma di giustizialismo. Siamo convinti che appurare l'esistenza o no del *fumus persecutionis* non debba comportare da parte del Senato una valutazione nel merito degli elementi probatori, anche se ciò non ci impedisce di sottolineare come il voto cui è chiamata oggi quest'Aula non sia in alcun modo paragonabile ad un'altra importante decisione richiesta contemporaneamente alla Camera dei deputati. *(Commenti dal Gruppo PdL)*. Ben altri sono i personaggi coinvolti, ben altri i reati contestati! Preso atto, infine, delle conclusioni della Giunta, che ha ritenuto opportuna la decisione di sottoporre la di una relazione informativa, ci limitiamo dunque a rilevare che non sembra sussistere alcun *fumus persecutionis* e ad escluderlo, quindi, ai danni del senatore Tedesco. Ne consegue direttamente il nostro accoglimento della domanda di arresti domiciliari formulata dall'autorità giudiziaria. Voglio infine ribadire il nostro augurio sincero al collega Tedesco perché possa dimostrare al più presto la sua totale estraneità ai fatti, nell'auspicio che la magistratura possa operare in tempi brevi con la massima serenità ed efficienza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci apprestiamo a decidere se autorizzare gli arresti domiciliari di Alberto Tedesco, senatore candidato al Senato in Puglia dal Partito Democratico, che ha fatto parte del Gruppo del Partito Democratico fino a febbraio di quest'anno e siede ancora oggi nei suoi banchi. Ci apprestiamo a decidere in ordine alla prerogativa più importante della funzione parlamentare, che è quella della inviolabilità personale di un senatore, e dico subito che noi vogliamo evitare che la prerogativa parlamentare della tutela della libertà personale di un parlamentare indagato si possa trasformare in un odioso privilegio. Ecco perché per noi la concessione dell'arresto di un parlamentare deve essere negata solo se c'è il sospetto di una volontà persecutoria, e dobbiamo accertare se dietro quell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP di Bari, poi trasformata in arresti domiciliari dal tribunale del riesame di Bari, e dietro le imputazioni formulate dalla procura di Bari si celi una persecuzione contro il senatore Tedesco. i capi di imputazione, che sono stati elencati prima, sono per gravissimi delitti contro la pubblica amministrazione, che sono stati contestati nell'ambito di un'indagine che è stata avviata dal 2007 dalla procura di Bari, nella quale, com'è stato detto, risultava coinvolto anche Nicola Vendola, detto Nichi. Dico anche che non condividiamo e non assecondiamo la tendenza a sostituire una giustizia sommaria alla giustizia a cognizione piena, a privilegiare il processo mediatico, perché è l'unico celebrato in tempi ragionevoli, rispetto invece al giusto processo previsto dall'articolo 111 della Costituzione. La giustizia perfetta non esiste? però, o dovrebbe esistere, una giustizia sollecita e responsabile, e questo per tutti: per i parlamentari e per tutti i cittadini di questo Paese. Dopo il verdetto definitivo si va in carcere per espiare una pena, ma la carcerazione preventiva, in assenza di un processo giusto e di una condanna definitiva, la detenzione prima del processo deve essere una eccezione. Nel pendolo di 19 riforme della custodia cautelare in 35 anni non siamo ancora riusciti ad evitare che la custodia cautelare in corso di processo sia la norma e non già invece un'eccezione. E non accettiamo nemmeno lezioni di giustizialismo, di antipolitica qualunquistica: due senatori di questa legislatura sono in carcere, e noi abbiamo già in Giunta e in Aula dimostrato di saper rispettare il lavoro della magistratura. E in uno Stato democratico occorre anche considerare l'interesse dell'indipendenza del Parlamento, evitando che ne venga alterata l'integrità della composizione come risulta dal voto democratico dei cittadini da iniziative della magistratura, che talvolta si rivelano del tutto infondate. Il quadro indiziario che emerge dalle enorme mole di atti d'indagine ci riporta comunque ad uno scenario inquietante. Nella sentenza del tribunale del riesame si riporta un'affermazione di un primario di ortopedia, tale dottor Canfora, che nel dicembre 2001 dichiara che bisogna vedersela con Alberto Tedesco per il ginocchio e con Salvatore Mazzaracchio, allora assessore regionale alla sanità, per l'anca, così testualmente dicendo: «una ripartizione delle sfere di influenza dei politici nella sanità pugliese, non già in funzione dello schieramento di appartenenza o della carica rivestita, ma addirittura in relazione alla parte anatomica in cui impiantare le protesi». Altro che Nenni, senatore Tedesco! Il consigliere regionale Tedesco, che nel 2001 si occupava di ginocchia e che agiva in maniera spregiudicata sul mercato dei prodotti sanitari e delle protesi, legato da rapporti d'affari con Giampaolo Tarantini, diventa nel 2005, grazie a Nichi Vendola, potente assessore alla sanità della Puglia, e nel 2008 senatore, grazie all'amicizia con il gruppo Columella di Altamura (riporto quello che è scritto nel provvedimento dell'aprile 2011 e grazie all'amicizia con il senatore uscente Donato Piglionica, il quale, dice il tribunale del riesame, ha contatti diretti con la senatrice Finocchiaro. I pubblici ministeri, prima, e il GIP, poi, descrivono un sistema sanitario pugliese marcio, di stampo clientelare, basato su una rete delinquenziale, su un sodalizio criminoso e su un sistema di lottizzazione politica sistematica delle cariche e degli appalti anche per interessi elettorali.

L'intercettazione telefonica fra Tedesco e Vendola - che ovviamente nessun giornale ha riportato - fa capire che Vendola conosceva bene i meccanismi di questo sodalizio criminoso e di questa sistematica Le dichiarazioni dell'indagata Lea Cosentino, ex direttore generale dell'ASL di Bari, nell'interrogatorio del luglio 2009, raccontano le sue preoccupazioni sulle infiltrazioni mafiose, sull'appalto per i rifiuti ospedalieri e sulla società Tradeco di Columella, esternate al presidente Vendola. Ovviamente la gara viene vinta dalla Tradeco, nonostante Vendola fosse perfettamente informato dalla Cosentino delle infiltrazioni mafiose. Vendola, astro nascente di Terlizzi, andava salvato, e così è stato; Tedesco doveva essere gettato al macero.

però, che non è persecutorio. Noi rimaniamo sempre basiti di fronte a queste definizioni. La procura e il GIP archiviano il caso di Vendola, presidente della Regione, ed invece adottano una posizione differente per un assessore. Dobbiamo anche chiederci se i reati contestati siano gravi. Sapete che esiste una prassi parlamentare al riguardo. Per il caso Margiotta, deputato del Partito Democratico, nel dicembre 2008

e sono sicuramente meritevoli di considerazione ai fini dell'arresto di un parlamentare. Dobbiamo decidere anche sulla base del contesto politico di oggi, tenendo conto delle numerose ed insistenti dichiarazioni del senatore Tedesco, rese anche oggi in Aula, e soprattutto delle dichiarazioni degli esponenti del suo partito, il Partito Democratico, con cui affermano di voler concedere l'autorizzazione all'arresto non essendoci ostacoli né giuridici né politici (così dichiara l'autorevole collega Casson).

Tedesco ci ha detto: «Non posso accettare che il Senato mi salvi. Voglio camminare a testa alta e voglio che la mia famiglia cammini a testa alta. Non potrei camminare fra la gente che dice che Tedesco è stato salvato dal Senato». dal Senato». Ci siamo chiesti perché non rivalutare l'istituto delle dimissioni, senatore Tedesco, e perché non evitare questo imbarazzo alle istituzioni parlamentari: se lei voleva camminare a testa alta, febbraio 2011 si sarebbe potuto dimettere in quest'Aula, noi avremmo accettato le sue dimissioni e oggi avremmo evitato questa situazione.

Concludo dicendo che, se i compagni di viaggio del senatore Tedesco, i furbetti del quartierino pugliese, coloro che lo hanno candidato al Senato ben conoscendo le indagini a suo carico, ne chiedono oggi l'arresto,

ringrazio, signor Presidente. questa mattina - lo dico a mo' di premessa - abbiamo assistito ad un inopinato dibattito in questa nostra Aula circa l'iscrizione all'ordine del giorno, anzitutto della 1a Commissione, dei disegni di legge costituzionale miranti a ridurre il numero dei parlamentari. Abbiamo assistito, anzi, ad una sorta di compiaciuta gara al rilancio su tali proposte, come se la credibilità della quota di classe dirigente nazionale impegnata in politica possa riprendere slancio da un semplice taglio di posti nelle due Aule parlamentari. Capisco che questo dipenda dal clima ormai irrespirabile intorno alla politica, ai suoi costi e ai suoi rischi: basti l'odierna rassegna stampa del Senato per farci capire il livello di accerchiamento. In questo senso, cercare di porre dei punti fermi di serietà, di garanzia di sobrietà, di conferma di impegno di servizio alla cosa pubblica costituisce impresa improba. Credo, tuttavia, che lasciare travolgere le istituzioni parlamentari nella sola polemica, anzi fomentarla per temporanei e - se posso dire - effimeri successi di parte, sia esercizio poco decoroso e poco confacente alle funzioni e al ruolo che, magari non degnamente, esercitiamo per un periodo della nostra vita. Quanto al di là di pressioni di opinione pubblica o giornalistica, è buona cosa anzitutto ripercorrere i precedenti. A questo, proposito non mi pare - ma lo ha già sottolineato il senatore Li Gotti

D'altro lato, non credo si possa conseguentemente utilizzare il caso e la persona per salvare l'immagine di quella che gergalmente è definita casta, sacrificando il singolo sull'altare dell'immediatezza della comunicazione. Credo possiamo concordemente confermare la assoluta adesione ai principi della legalità quali fondamenti dell'azione politico‑amministrativa, talché nessuno dubita che la magistratura debba assolutamente perseguire i reati e chi li compie, senza alcuna remora. Credo, altresì, che non possiamo non esprimere un giudizio politico di estrema perplessità per le modalità gestionali della sanità pugliese. Oggi ci viene chiesto di autorizzare l'arresto, nelle forme indicate, con riferimento ai rischi che lo *status* di senatore dell'indagato può far insorgere per condizionamenti e reiterazioni vari... Colleghi, capisco che vi sia un po' di stanchezza, però stiamo discutendo di temi estremamente delicati, che riguardano la libertà delle persone, in particolar modo di un componente di quest'Assemblea. quindi, tutti i colleghi a una maggiore compostezza, e chi non è interessato ad ascoltare il senatore Molinari è pregato di lasciare l'Aula. Prego, senatore Molinari. Sotto questo profilo, non può non colpire la nostra attenzione la descrizione che negli atti depositati viene fatta dal giudice richiedente circa, appunto, il nostro *status* di senatori della Repubblica. Se al cognome del senatore interessato sostituissimo il nostro, resteremmo colpiti dall'idea esplicita di una nostra automatica propensione alla occupazione, anziché all'esercizio, del potere parlamentare. Descrizione questa che nella sua oggettiva assolutezza non credo possiamo proprio accettare. Peraltro e purtuttavia, nella convinzione che non possano esistere correlazioni di alcun tipo, né come tipologie penali e men che meno per modeste questioni pseudo-politiche fra il dibattito qui in corso e quello ora in corso presso la Camera dei deputati, senza entrare nel merito dei reati contestati (perché non siamo chiamati a questo), per i quali è auspicabile che la magistratura proceda ad ogni chiarimento, l'orientamento del Gruppo al quale do voce è che non possiamo non prendere atto della richiesta motivatamente espressa dall'interessato, che intendiamo rispettare nell'espressione Signor Presidente, onorevoli colleghi, se non fossi ormai abituata, se non avessi un lungo allenamento

essermi confusa. Una certa confusione, infatti, mi pare che stia segnando questa discussione. Da parte dei colleghi della maggioranza, in particolare del PdL, i ad ogni piè sospinto rivendicano la propria appartenenza all'unico partito che abbia una concezione garantista

Il senatore Tedesco ha citato Pietro Nenni; io citerei Totò, e quel «più oltre» che deve sovvenire nei momenti di grande difficoltà, quando improvvisamente il terreno ti manca sotto i i piedi e ti inoltri in una terra che non ti è conosciuta, quella della dignità sobria che oggi abbiamo ascoltato nell'intervento del senatore Tedesco: la sobrietà nel misurare il pericolo per le istituzioni e la loro autorevolezza, quella misura con la quale si dice: «Per quello che posso fare non contribuirò alla ruina», hanno tracciato un campo sul quale - ho capito - scivolate. E non bastano neanche le acrobazie del senatore Mazzatorta, il quale tra l'altro ha fatto un riferimento a me, che non ho colto esattamente nei contenuti, ma che nell'intervento mi è sembrato offensivo, per cui chiedo il giurì d'onore, Presidente.

Una diffidenza che vedo soprattutto nei confronti della rappresentanza, quasi a ripercorrere un filone di pensiero politico che fu della Destra storica, nella quale l'istanza quale l'istanza autoritaria e populista faceva sacrificio delle ragioni della rappresentanza, viste addirittura come impedimento, come fattore di demodernizzazione - al contrario di quanto ciascuno di noi ritiene in quest'Aula - di un Paese e delle sue forme democratiche.

Ma perché ti stai irritando? Non sto parlando con te, sto svolgendo un ragionamento al quale sto cercando di associare tutti. Un Parlamento tanto meno autorevole è tanto più comodo a chi alle ragioni della rappresentanza non annette il valore che tutti noi vi annettiamo.

E non è la paura che deve muoverci, né farci asserragliare, né farci assolutamente condiscendenti o assecondanti. Qualunque critica, anche le più becere, anche le meno colte, anche le più venate da un'irritazione e da una rabbia che non ha ragioni,

trasparenza, che qui assumiamo. Ed è questa la ragione per la quale Alberto Tedesco chiede che venga concessa l'autorizzazione agli arresti, ed è la ragione per la quale il nostro Gruppo così voterà.

una ragione semplice, collega Asciutti. Non capisco perché a un qualunque magistrato della Repubblica viene chiesto il coraggio di pronunciare pubblicamente in aula una sentenza o di firmare un provvedimento, e a un parlamentare della Repubblica bisogna dare l'ombra del voto segreto.

Qualunque sarà la determinazione che verrà assunta oggi in quest'Aula sulla richiesta di custodia cautelare nei confronti del senatore Tedesco, anche nel caso in cui, come noi auspichiamo, tale richiesta sarà respinta, non stiamo affermando che nella sanità pugliese in questi anni non sia successo niente. Non stiamo cancellando con un colpo di spugna una storia di clientele e clientelismi, di nomine, appalti e inopportune commistioni che sul piano politico ci sentiamo di dover stigmatizzare, come ha fatto poco fa il collega Amoruso. Dirò di più, signor Presidente: se oggi il PdL può permettersi di difendere il Parlamento e dire «no» all'arresto del senatore Tedesco senza timore che questo passi per un'assoluzione politica, è perché il centrodestra non ha aspettato che intervenisse la magistratura per denunciare pubblicamente una gestione della sanità opaca, come fabbrica di voti e serbatoio di affari, da parter del centrosinistra, dell'ex assessore Tedesco e dello stesso presidente Vendola. Il collega Saccomanno potrebbe testimoniare le lunghe sedute del Consiglio regionale della Puglia, nella passata legislatura, spese a far presente al presidente Vendola quanto difficilmente conciliabili fossero gli interessi della famiglia Tedesco in campo sanitario con il ruolo di assessore nello stesso settore. Cosa accadeva nel sistema della sanità pugliese lo sapeva, dunque, anche il presidente Vendola, che a suo tempo si presentò in Consiglio regionale a difendere il suo assessore, salvo poi vestire i panni del moralizzatore alle prime avvisaglie di un interessamento dell'autorità giudiziaria, come se questo bastasse a cancellare le responsabilità politiche. E in tempi assai lontani, prima ancora che la sinistra conquistasse il Governo della Regione Puglia, la stessa procura di Bari, quella della precedente gestione per intenderci, sapeva in che modo l'allora consigliere Alberto Tedesco cercasse di favorire affari che gli stavano a cuore. Ma mentre concentrava straordinarie attenzioni su Raffaele Fitto il senatore Li Gotti che ha letto i documenti lo sa meglio di me - quella procura assolveva Tedesco e anzi non lo indagava proprio. A rilevarlo, colleghi, non siamo noi, ma gli stessi magistrati. Basta leggere, ad esempio, il provvedimento del tribunale del riesame sul caso del quale ci stiamo occupando. Ma non è questo il centro del problema. Noi stiamo per votare la richiesta di arresto preventivo di un parlamentare. Sull'uso della custodia cautelare nel nostro Paese auspichiamo prima o poi un dibattito *ad hoc*. In questa sede vale, però, la pena ricordare che nella nostra procedura penale le misure cautelari servono a impedire la fuga, l'inquinamento delle prove, la reiterazione del reato, ed è prassi che il Parlamento valuti anche questi aspetti e non solo l'eventualità di un *fumus*. Le misure cautelari hanno dunque un senso se sono immediate e in qualche modo "a sorpresa". Se l'indagato sa con largo anticipo della richiesta di arresto pendente nei suoi confronti, com'è inevitabile che sia nel caso di un parlamentare a causa delle procedure previste, avrebbe tutto il tempo di scappare, inquinare le prove o reiterare il reato. La vicenda di Toni Negri in tal senso è eloquente. Né quest'Aula può accedere alla tesi per cui Alberto Tedesco, pur avendo cessato ogni carica nella Regione Puglia, potrebbe reiterare il reato in quanto senatore, quasi che la qualifica di parlamentare fosse in qualche modo criminogena. Presidente Finocchiaro, non si difendono così il nostro onore e le nostre istituzioni! L'idea dell'arresto preventivo di un parlamentare, insomma, ci convince poco già sul piano della logica. Ma al di là di questa c'è una ragione più profonda che investe il fondamento stesso delle nostre istituzioni. Senatore Tedesco, mi rivolgo a lei con la dura lealtà che si deve a un avversario politico in un momento come questo. Lei aveva chiesto nei suoi interventi pubblici e in Giunta che il Senato che il Senato riconoscesse l'esistenza di un *fumus* nei suoi confronti o, in alternativa, autorizzasse il suo arresto, e ancora oggi chiede al Senato di farla arrestare. Noi che ragioniamo dal punto di vista delle istituzioni la pensiamo esattamente al contrario. Quest'Aula non la può assolvere perché non è un tribunale. A giudicarla penalmente ci penseranno i magistrati. E a nostro avviso, lei non è un perseguitato. Ma noi possiamo difendere le sue prerogative, perché difendendo le sue prerogative difendiamo il Parlamento, le istituzioni e lo Stato. E lo facciamo da avversari, esprimendo il giudizio politico più pesante sul suo operato. Perché noi sappiamo distinguere. Senatore Tedesco, se invece lei ritiene di voler andare incontro alla giustizia - mi dispiace, senatrice Finocchiaro, Totò non c'entra niente

ma non può pretendere da noi l'abbattimento di quell'ultimo residuo contrappeso nel rapporto tra giustizia e istituzioni rappresentative della sovranità popolare. Si dimetta, senatore Tedesco, e consenta a chi era in lista dopo di lei di prendere il suo posto e garantire il *plenum* dell'Aula, così come lei si è trovato "casualmente" a sostituire il senatore De Castro dopo le ultime elezioni europee. *(Applausi dai lei lo sa bene, perché viene dalla sua terra. C'è chi, prima del senatore Tedesco, da questi stessi scranni è andato incontro alla galera, ma non ha preteso che la sua scelta personale gravasse sulle istituzioni. Lei può fare altrettanto, senatore Oggi abbiamo letto un'intervista nella quale lei sostiene che le sue dimissioni sarebbero un *vulnus* nei confronti del Senato. No, senatore Tedesco, ancora una volta è vero il contrario: il vero *vulnus* nei confronti del Parlamento sarebbe dire sì alla richiesta di arresto. Colleghi della sinistra, sappiamo bene che fuori da queste mura già si preparano nuovi roghi, nuove pire - ha fatto riferimento anche ad esse, senatore Tedesco ma se ci troviamo qui dentro siamo tenuti anche al coraggio di decidere non sulla base della convenienza politica di un momento, ma di princìpi che valgono per gli amici e per gli avversari, per chi è innocente e anche per chi sarà, forse, riconosciuto colpevole. L'antipolitica non si può sfamare, collega Finocchiaro, dandole in pasto le istituzioni o consegnando alla magistratura la facoltà di intaccare l'integrità del *plenum* delle Camere, e dunque determinare l'esistenza o meno delle maggioranze e la sopravvivenza dei Governi. Ai tempi del Governo Prodi, con un solo voto di scarto in Senato, ci sarebbe voluto davvero poco perché ciò accadesse. Ai nostri avversari diciamo dunque: fermatevi, pensateci bene. Non consentite che a trionfare sia l'antiparlamentarismo travestito da politicamente corretto, altrimenti da qui a breve la politica, la politica di tutti, e le istituzioni, quelle di tutti, ne potrebbero restare travolte. Gli eventi del insegnare qualcosa anche a voi. I partiti hanno a disposizione molti strumenti per sanzionare politicamente comportamenti che si ritengono scorretti. Esistono le sospensioni, le espulsioni, la possibilità di migliorare la qualità della classe dirigente e della rappresentanza Ma questa responsabilità, che è politica, non la si può scaricare sulle spalle delle istituzioni. E se proprio non ce l'avete il coraggio di fondare il vostro parlamentarismo su principi solidi, ancorché qualche volta impopolari; se proprio non ce la fate a resistere al richiamo dell'antipolitica ed a sopportare il suo giudizio sommario, vorrà dire che ci faremo carico noi di difendere le istituzioni. E lo faremo! Lo faremo anche in nome di una parte della vostra tradizione. Andate a leggere le pagine di Umberto Terracini o di Fausto Gullo. Senatore Tedesco, le consiglio una citazione di Pietro Nenni, ancora attualissima: non c'è nessun puro che prima o poi non venga epurato da qualcuno più puro di lui. ha chiesto a quest'Aula di essere assolto o di essere arrestato. Io chiedo al Gruppo del PdL e a tutta l'Assemblea, a voto segreto, perché non riconoscere uno spazio alla coscienza quando è in gioco la libertà personale significherebbe essere a un passo dalle pratiche dei regimi totalitari *(Applausi parlamentari *­*- di non assolverla, ma di non acconsentire a un arresto che sarebbe ingiusto per lei, grave per le istituzioni parlamentari, offensivo per ciò che tutti noi rappresentiamo, perché annullerebbe il giudizio politico facendolo coincidere con il giudizio penale, per giunta con rito abbreviato. *(Vivi

Presidente e colleghi, credo che il dibattito che questa sera si è svolto nell'Aula del Senato abbia dato una volta di più, se possibile, la dimostrazione di quanto sia urgente nel nostro Paese affrontare la riforma della giustizia.

che è quello - ritengo - di evitare nel modo più assoluto di decidere sotto la pressione della piazza e dell'antipolitica. Credo che noi siamo qui non per mandare la gente in galera. Siamo qui per difendere l'istituzione Parlamento attraverso un lavoro serio, trasparente, assiduo, costante, onesto. Siamo qui soprattutto per difendere l'interesse generale del popolo italiano. Siamo qui per difendere la democrazia, che è costata tante vite e tanto sacrificio. Siamo qui soprattutto, Presidente, per dire a testa alta, tutto quel fango che ci viene quotidianamente riversato addosso, che è ora di finirla! È ora di finirla, assumendosi la responsabilità di dirlo, anche andando incontro ad una impopolarità generalizzata: non me ne può importare di meno, meno, è ora di finirla e di dire basta a tutto questo! Cari colleghi, oggi il cappio si può stringere attorno ad una gola; domani si potrà stringere attorno ad altre gole e poi si stringe attorno a tutti. Ed è vero, senatrice Finocchiaro, che se andiamo avanti di questo passo rimetteremo in piedi i podestà ed i dittatori,

se è vero com'è vero - lui lo ha detto e non posso assolutamente dubitarne - che il procuratore di Bari un mese fa ha detto che le indagini erano chiuse, allora, collega Li Gotti - lo dico a lei che ha più esperienza e più cultura specifica nel campo -

un reato? Se le indagini sono chiuse, è impossibile. C'è una contraddizione di fatto. Quindi, per rispetto del Parlamento, di quelle prerogative parlamentari alle quali i nostri Padri costituenti ci hanno legato con grande saggezza,

nel momento in cui si è candidato, all'epoca, un ex assessore per evitare che andasse in galera e, oggi, si fa moralismo cercando di evitare che quell'assessore vada in galera. È una contraddizione di una pesantezza tale che mi porta a dire: un conto è il moralismo, un conto è il cinismo. Voi state compiendo un atto di cinismo, non un atto di moralismo!

secondo la senatrice Finocchiaro, farlo con voto palese. Se c'è una valutazione che deve essere fatta a scrutinio segreto è proprio questa.

Tuttavia devo osservare che la sua risposta copre il suo comportamento in Aula, cioè il suo diritto a portare in Aula la relazione del senatore Li Gotti, ma non copre il comportamento del Presidente della Giunta delle elezioni.

Nella stessa circostanza e nella stessa situazione, l'omologo del senatore Follini alla Camera ha messo in votazione la relazione, all'ultimo momento, per consentire all'Aula di esprimersi. Lui non lo ha fatto. Perciò il presidente della Giunta

Lei ha cercato di esonerare dalla sua responsabilità un autorevole dirigente del suo partito; ne prendo atto. Sicuramente quell'autorevole dirigente non l'avrà convinta.

però, senatore Tedesco, ho un problema con lei, perché lei ha detto: primo, i fatti che mi sono

Dopodiché, lei ha aggiunto...

pesi diversi da parte di giudici diversi, oppure il fatto che alla chiusura delle indagini non sia seguito il processo - dopo averci detto: «c'è un *fumus*, io sono innocente» lei ha aggiunto: «siccome sono innocente, cari amici, arrestatemi». Questo è esattamente ciò che è scritto in quelle pagine buie del romanzo «Buio a mezzogiorno».

in questione fa riferimento esplicito al caso in cui non ci sia una decisione della Giunta, perché afferma che, in difetto, si procede in una certa maniera. Nel nostro caso, non era stata approvata la relazione del senatore Balboni, quindi non c'era nessuna relazione di minoranza e pertanto correttamente è stato delegato un altro senatore. PRESIDENTE. Senatore Casson, il tema è stato abbondantemente dibattuto e poi la Presidenza si è assunta una responsabilità interpretativa.

ai sensi dell'articolo 135, comma 10, del Regolamento, coloro i quali sono favorevoli a concedere l'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare agli arresti domiciliari voteranno sì, premendo il tasto verde; coloro che invece sono contrari alla concessione all'autorizzazione voteranno no, premendo il tasto rosso; coloro che intendono astenersi, si comporteranno di conseguenza, premendo il tasto bianco.

sono autorizzate a convocarsi al termine della seduta odierna al fine di concludere l'esame del decreto-legge recante la proroga delle missioni internazionali. La discussione in Aula, conformemente a quanto stabilito dal calendario dei lavori approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo di ieri, avrà luogo nella seduta antimeridiana di domani, secondo i tempi ripartiti. **Mozioni,